con efficacia immediata, che è vietato l'accesso a tutte le sedi del Senato al parlamentare che non esibisce il *green pass.* Laddove si verifichi un accesso non consentito, viene irrogata immediatamente la sanzione di divieto di accesso a tutte le sedi del Senato e di interdizione ai lavori parlamentari per dieci giorni. *(Applausi)*. Per tali ragioni il Consiglio dispone, con efficacia immediata, l'irrogazione della sanzione sopra descritta alla senatrice Bianca Laura Granato. L'ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro dell'interno sui gravi fatti accaduti a Roma il 9 ottobre scorso in occasione della manifestazione svoltasi presso Piazza del Popolo».

rivolgo un sentito ringraziamento a questa Assemblea per avermi offerto l'opportunità di svolgere un'informativa sui gravi disordini verificatisi in occasione della manifestazione contro l'introduzione del *green pass*, svoltasi a Roma il 9 ottobre scorso. Nella seduta del *question time* di mercoledì scorso alla Camera dei deputati, in un'interrogazione a me rivolta erano stati chiesti chiarimenti riguardo a quella manifestazione, con specifico riferimento alla circostanza che vi fossero presenti esponenti di Forza Nuova. I tempi estremamente contingentati, che connotano lo specifico strumento di sindacato ispettivo, mi hanno consentito di trattare solo molto parzialmente un tema - quello dell'ordine pubblico e delle infiltrazioni criminali nelle manifestazioni di protesta correlate alle misure governative di contenimento della pandemia che merita certamente una più ampia e approfondita disamina. Per questo motivo ho dato immediatamente la mia disponibilità a riferire anche sui successivi fatti di Milano e Trieste, in considerazione del fatto che essi si inquadrano nello stesso contesto, essendo collegati alle medesime forme di protesta. Prima di entrare nel merito degli episodi di violenza accaduti a Roma, riguardo ai quali rinnovo la mia solidarietà alla CGIL e la mia vicinanza alle Forze di polizia è questa l'occasione per offrire a entrambi i rami del Parlamento una complessiva visione di come è stata impostata, in questi due anni circa di pandemia, la politica dell'ordine pubblico. È apparso subito chiaro che le restrizioni alla mobilità e i sacrifici imposti dalle misure anti contagio potessero suscitare uno stato di insofferenza diffusa, anche esasperato dalle ricadute di natura economica e occupazionale derivanti dal blocco o dal rallentamento delle attività produttive e commerciali. In questo periodo è stata messa alla prova la capacità di resilienza dell'Italia, che ha reagito in maniera seria e composta, attingendo al patrimonio delle proprie migliori qualità morali e civili. La tenuta del Paese, anche dal punto di vista dell'ordine pubblico, deve molto all'elevato senso di responsabilità con cui è stata vissuta e si sta vivendo questa difficilissima prova. Non sono mancate tuttavia nel 2020, e anche nel corso di quest'anno, manifestazioni di acceso dissenso, indirizzatesi verso le diverse misure che il Governo ha di volta in volta adottato e calibrato in ragione dell'evolversi della curva pandemica ai fini della limitazione del contagio. È risultato evidente il rischio che la protesta e il malcontento sociale, innescati dagli effetti depressivi della pandemia, potessero essere oggetto di strumentali intrusioni da parte di frange eversive di vario orientamento politico e ideologico, interessate a rilanciare progettualità conflittuali e istanze destabilizzanti, anche canalizzando forme spontanee e trasversali di ribellismo, rimaste finora prive di una regia unitaria. La consapevolezza di questo complesso scenario ha portato a sensibilizzare, con una mia direttiva dell'aprile del 2020, la rete delle prefetture per monitorare attentamente segnali di criticità e prevenire possibili derive violente in grado di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica. Con successive indicazioni operative non si è mancato di raccomandare il ricorso a modalità di gestione della piazza improntate al più grande equilibrio, contemperando il diritto a esprimere pacificamente il dissenso con la necessità di salvaguardare l'ordinata convivenza civile. Non sfugge peraltro come una diversa strategia, che non rapporti l'impiego della forza a questa esigenza di equilibrio, presenti il pericolo di offrire speciosi argomenti a narrazioni antisistema, in grado a loro volta di coagulare e dare copertura alle spinte più decisamente oltranziste. Vorrei affidare questa mia analisi all'evidenza dei fatti. Dal febbraio 2020 al 18 ottobre 2021 si sono tenute in Italia 5.769 manifestazioni di protesta contro i provvedimenti governativi di contenimento del virus; più della metà (precisamente 3.668) si sono svolte nel 2021 e di queste 1.526, tenutesi tra il 22 luglio e il 18 ottobre di quest'anno, hanno riguardato la contestazione al *green pass.* Nello stesso periodo 22 luglio - 18 ottobre 2021, lo sforzo di contenimento delle contestazioni di piazza alle certificazioni verdi ha portato all'assegnazione di 17.470 unità delle forze mobili di polizia alle autorità di pubblica sicurezza. La percentuale delle iniziative di protesta che in tale arco tempo temporale hanno registrato episodi di rilievo sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica si attesta al 3,4 per cento, riguardando soltanto 52 manifestazioni. Il principio per il quale l'ordine pubblico in piazza deve essere gestito sempre con equilibrio lo ritengo un elemento cardine della democrazia. È un principio a cui le forze di polizia si stanno attenendo non da oggi e che risulta imprescindibile se non vogliamo che tra chi manifesta e chi difende il diritto a manifestare si crei una pericolosa cortina di ostilità o diffidenza. Passo ora a riferire sulla manifestazione del 9 ottobre, che ha rappresentato senza dubbio l'evento più gravemente critico nell'ambito della mobilitazione nazionale contro il *green pass.* Premetto che nell'immediatezza dei fatti ho chiesto al Capo della polizia e direttore generale della pubblica sicurezza una dettagliata ricostruzione delle evidenti criticità che - occorre riconoscerlo - hanno contrassegnato la gestione dell'ordine pubblico di quelle ore. È palese che non si sia riusciti a contenere tutti i propositi criminali da cui era mossa la parte violenta dei manifestanti, specie quella istigata dagli elementi più politicizzati e in conseguenza dei quali vi è stata una grave turbativa dell'ordine pubblico. Il successivo 13 ottobre, nella riunione del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica convocata per le misure relative al G20 di fine mese, alla quale hanno partecipato i vertici degli organismi di *intelligence,* il prefetto, il questore di Roma, i rappresentanti del Ministero della difesa, nonché ovviamente i vertici delle Forze di polizia, ho sottolineato l'esigenza che il *deficit* di sicurezza determinato da una situazione che ha superato ogni ragionevole previsione non debba più ripetersi; ciò soprattutto in considerazione della delicata fase che si sta attraversando e per il combinato effetto di diversi fronti: dall'applicazione del *green pass* alle crisi aziendali, fino ai delicati riflessi della protesta dei portuali e degli autotrasportatori sulla logistica delle merci. Ci attende un periodo ancora molto impegnativo che, peraltro, vedrà a fine ottobre - come ho detto - lo svolgimento del vertice dei Paesi del G20. È da considerare prezioso in questa fase l'apporto informativo volto a focalizzare ogni possibile fonte di rischio e i pericoli maggiori, nonché a indirizzare le stesse attività di mediazione che pure hanno dimostrato in varie occasioni la loro efficacia nell'abbassare la tensione e nel decongestionare la piazza. La mia informativa si baserà sugli elementi fornitimi dal Capo della polizia e si soffermerà su alcuni interrogativi che hanno caratterizzato il dibattito politico e mediatico sviluppatosi nei giorni successivi. L'iniziativa di Roma ha visto - come è noto - una partecipazione composita e assai eterogenea. Infatti, accanto a esponenti di gruppi e movimenti politici appartenenti sia alla destra radicale che alla galassia della sinistra antagonista e alla componente anarchica, vi hanno preso parte rappresentanti di categorie economiche e anche semplici cittadini intenzionati a contestare le misure di contenimento del Covid, ritenendole l'espressione di un disegno autoritario volto ad affermare la cosiddetta dittatura sanitaria. Un primo aspetto da chiarire attiene all'adeguatezza del dispositivo di ordine pubblico approntato dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza in rapporto all'elevato numero dei manifestanti, tra le 10.000 e le 12.000 persone riversatesi a Piazza del Popolo e nelle altre strade del centro di Roma. È stata rimarcata, infatti, una sproporzione tra i due elementi in raffronto, al punto da interrogarsi se ci sia stata o meno una sottovalutazione dell'evento, dipesa anche da una carenza del circuito informativo. Chiarisco che gli organizzatori della manifestazione, nel darne il prescritto preavviso alle autorità di pubblica sicurezza, avevano indicato in 1.000 persone il numero orientativo dei partecipanti. Avuto però riguardo al fatto che l'iniziativa si sarebbe tenuta appena una settimana prima dell'introduzione dell'obbligo del *green pass*, le stesse autorità hanno ritenuto che l'affluenza effettiva si andasse invece ad attestare tra le 3.000 e le 4.000 unità. Coerentemente a tale previsione, la forza pubblica messa a disposizione della questura di Roma era di 590 elementi, a cui si andavano a sommare 250 operatori della forza territoriale appartenenti anche all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza. Pertanto, il complessivo dispositivo poteva contare su 840 unità effettive da ritenersi pienamente adeguato in termini di proporzionalità rispetto alle stime previsionali. Non erano poi mancati, nella stessa mattinata del 9 ottobre, diffusi controlli sui caselli autostradali e agli snodi della mobilità cittadina, che avevano portato all'individuazione e identificazione di poco meno di un migliaio di manifestanti, provenienti prevalentemente dalle Regioni del Nord Italia, segnalando un flusso in arrivo in linea con quello preventivato. Anche la manifestazione di Piazza del Popolo, al pari delle precedenti contro il *green pass* e le altro no vax e no mask, era stata preannunciata da un'intensa campagna informativa lanciata sui più diffusi *social network.* Tuttavia, diversamente dalle precedenti manifestazioni, che pur sostenute dallo stesso ampio *battage* avevano fatto registrare presenze assai contenute e ben distanti dagli enfatici richiami degli organizzatori, quella del 9 ottobre inaspettatamente ha attirato un numero di partecipanti più che triplicato rispetto a quello previsto, addensatosi in poco tempo in Piazza del Popolo. Peraltro, l'assenza di elementi informativi da qualsiasi fonte non consentiva di prefigurare un indice di partecipazione così anomalo rispetto ai precedenti. Un altro aspetto critico attiene alla partecipazione di esponenti di Forza Nuova alla manifestazione del 9 ottobre. Tale presenza, che ha complessivamente raggiunto circa 200 unità, non fa che confermare l'acceso interesse di questa formazione, notoriamente appartenente all'area della destra radicale ed estremista, ad acquisire, attraverso l'adesione alla protesta, spazi di visibilità che ne accrescono il bacino di consenso. Gli esponenti di spicco di Forza Nuova che hanno preso parte alla manifestazione si sono poi evidenziati soprattutto nella fase degli scontri e durante l'assalto alla sede della CGIL, come dimostrano le misure cautelari disposte nei loro confronti. È stata al centro dell'attenzione la presenza in Piazza del Popolo di un noto esponente romano di Forza Nuova, Giuliano Castellino, vice segretario nazionale del movimento. Da più parti, infatti, si è chiesto come sia accaduto che un soggetto ben noto alle Forze dell'ordine per i suoi trascorsi delinquenziali, destinatario di un Daspo con divieto di partecipare alle manifestazioni sportive, nonché della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, si sia potuto recare a una manifestazione pubblica a cui ha preso parte attiva. Va chiarito che, secondo un rigoroso orientamento che tiene conto dei più recenti esiti della giurisprudenza nazionale e sovranazionale, ossia della CEDU e della Corte costituzionale in materia di misure di prevenzione, la facoltà di arresto della persona soggetta a sorveglianza speciale, disciplinata dall'articolo 75 del decreto legislativo n. 159 del 2011, viene ora correlata alla violazione di quelle prescrizioni che abbiano un contenuto determinato e specifico e che siano quindi compatibili con i principi costituzionali. Tale più stringente orientamento è stato oggetto di pregresse interlocuzioni con la magistratura requirente, con riguardo proprio all'applicazione nei riguardi del Castellino della generica prescrizione di non partecipare a manifestazioni pubbliche se non dopo averne dato preavviso alle autorità di pubblica sicurezza. In sostanza, solo la ricorrenza, nel pomeriggio del 9 ottobre, di altri validi motivi di legge ne ha poi potuto giustificare a titolo diverso l'arresto. È stato riportato da diversi servizi giornalistici che Giuliano Castellino, salito sul palco di Piazza del Popolo, ha indicato a tutti i manifestanti, con particolare violenza verbale, che di lì a poco si sarebbero diretti verso la sede della CGIL per assaltarla, sicché ci sarebbe stata una sorta di proclama di un disegno criminoso a cui non si sarebbe data un'adeguata risposta. Di qui una lettura politica che, utilizzando espressioni riecheggianti stagioni drammatiche della storia della Repubblica, tende ad accreditare la tesi secondo cui tale disegno sarebbe stato quasi assecondato, nella sua attuazione, dal comportamento delle Forze dell'ordine. Devo respingere fermamente questa lettura. *(Applausi)*. Essa, oltre a non tener conto del susseguirsi dei fatti, insinua il dubbio che le Forze di polizia, a cui dobbiamo la difesa delle istituzioni e il mantenimento della pace sociale, si prestino a essere strumento di oscure finalità politiche. È un'ingiusta accusa, che getta un'ombra inaccettabile sull'operato delle Forze dell'ordine, le quali nelle manifestazioni del 9 ottobre hanno pagato il tributo di ben 41 feriti, anche per fronteggiare i facinorosi intenzionati ad assaltare le sedi istituzionali. Si è poi anche adombrata l'ipotesi della possibile presenza in piazza di agenti infiltratisi tra i manifestanti. Sento di dover escludere anche questo inquietante retroscena. Nel dispositivo era prevista - come è normale - la presenza di agenti in borghese appartenenti alla Digos con compiti di osservazione, monitoraggio e anche mediazione con i manifestanti. Agli stessi compiti era addetto anche l'operatore di polizia che in abiti civili compare in alcune immagini diffuse sui *social* presente alle azioni di alcuni esagitati che intendevano provocare il ribaltamento di un furgone della polizia. In realtà, quell'operatore stava verificando che la forza scaricata sul mezzo non riuscisse effettivamente nell'intento. Si tratta dello stesso agente che più tardi, aggredito da un manifestante da lui arrestato

ha reagito in modo scomposto e per questo motivo si è autosegnalato ed ora la sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria. Ritornando alla figura e al ruolo di Giuliano Castellino, è importante precisare la tempistica dei suoi interventi dal palco di Piazza del Popolo, soprattutto rispetto a un altro punto critico che qui intendo approfondire, ossia l'assalto alla sede della CGIL. Dopo aver preso la parola una prima volta poco dopo le ore 15, senza fare alcun riferimento alla CGIL, Castellino riprende a parlare in pubblico alle ore ossia un quarto d'ora dopo che Luigi Aronica, altro esponente di Forza Nuova, facesse richiesta ai responsabili della sicurezza di consentire lo svolgimento di un corteo che, attraversando Villa Borghese, arrivasse fino alla confluenza con Corso d'Italia. Nei pressi della sede della CGIL i manifestanti, secondo la richiesta in quel frangente formulata, ma non autorizzata, si sarebbero soffermati - a loro dire - per scandire slogan di protesta e disapprovazione. È evidente, dunque, come l'intenzione dei manifestanti di dirigersi verso la sede sindacale non sia stata il frutto estemporaneo dell'incitamento di Castellino, ma fosse emersa già da prima, in quanto oggetto di una esplicita richiesta in corso di valutazione da parte delle autorità di polizia, le quali frattanto avevano invitato i manifestanti ad attendere, anche al fine di indicare loro percorsi e siti alternativi. Alle 16,45, senza che fosse stata accordata alcuna autorizzazione, un considerevole numero di dimostranti (circa 3.000) iniziava improvvisamente a muoversi in corteo verso Piazzale Flaminio, con l'intenzione di raggiungere Piazzale del Brasile. L'avanzata dei manifestanti è avvenuta in maniera impetuosa e alquanto disordinata, e per un breve momento è riuscita a superare gli stessi operatori di polizia. Ciò ha fatto sì che le Forze dell'ordine abbiano accusato una grave difficoltà di reazione, causata essenzialmente da una situazione venutasi ad accelerare in pochissimi minuti; nondimeno sono intervenute immediatamente per frenare la rapida avanzata del corteo, anche invitando i manifestanti a desistere e, allo stesso tempo, per predisporre la rimodulazione dei servizi al fine di approntare una barriera di contenimento in Piazzale del Brasile, alla confluenza con Corso d'Italia. In questa fase assolutamente dinamica i funzionari di polizia hanno avuto interlocuzioni anche con Castellino, il quale nel frattempo aveva raggiunto la testa del corteo; interlocuzioni che erano tuttavia esclusivamente funzionali a guadagnare tempo per il rischieramento del personale e dei mezzi. ore 17, in Piazzale del Brasile si sono schierate sei squadre dei reparti inquadrati, per un totale di 60 uomini, dirette da un funzionario della Polizia di Stato, mentre ulteriori due squadre, per complessive venti unità, andavano a posizionarsi nei pressi della sede della CGIL. Frattanto, un consistente dispositivo di contenimento veniva disposto verso Via del Tritone per fronteggiare il prevedibile e concomitante tentativo dei manifestanti di raggiungere le sedi istituzionali. Il numero esorbitante dei partecipanti al corteo e anche il loro impeto hanno tuttavia rappresentato una forza d'urto capace di superare lo sbarramento velocemente approntato a Piazzale del Brasile, così aprendo un varco ai manifestanti, dei quali circa 1.500 si dirigevano verso l'ingresso principale della CGIL, mentre gli altri defluivano verso Via Veneto, con il chiaro intento di arrivare a ridosso di Palazzo Chigi e Montecitorio. Durante questa turbolenta fase di scontro, caratterizzata da un'evidente sproporzione tra la massa di manifestanti e le Forze dell'ordine in campo impegnate a coprire vari fronti, è rimasto seriamente ferito, riportando la frattura di una costola, il funzionario di Polizia che comandava i nuclei in servizio. L'intervento delle Forze di polizia a difesa della sede della CGIL, pur avvenuto in un frangente di estrema concitazione, si è dispiegato almeno inizialmente in maniera tale da non evitare il prevalere dell'azione eversiva. È accaduto perciò che, grazie all'effrazione di una finestra laterale avvenuta alle 17,27, un piccolo gruppo di facinorosi sia riuscito a penetrare all'interno del pianoterra e, conseguentemente, a forzare la porta principale dell'ingresso, consentendo anche ad altri manifestanti, presenti all'esterno, l'accesso all'edificio. Questo è stato il momento più drammatico di quel sabato pomeriggio, che ha turbato fortemente l'opinione pubblica per la violenza dell'azione distruttiva e per lo sfregio alla democrazia che esso ha rappresentato; un momento durato otto angoscianti minuti e che ha avuto il suo apice dalle 17,32, quando i manifestanti irrompono nella sede sindacale, alle 17,35, allorché le Forze di polizia riprendono il pieno controllo della situazione e liberano i locali della CGIL, proteggendoli dalle possibili ulteriori pressioni dei manifestanti. I principali responsabili di questo vile assalto, in virtù dell'istituto della flagranza differita, sono stati tratti in arresto; si tratta di sei persone accusate di devastazione e saccheggio, istigazione a delinquere, danneggiamento, violazione di domicilio aggravata, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Tutte le persone arrestate sono ancora detenute in custodia cautelare. Le misure coercitive hanno raggiunto i due capi di Forza Nuova, Roberto Fiore e Giuliano Castellino, il loro sodale Luigi Aronica, Salvatore Lubrano, esponente di un'organizzazione della destra radicale, e Pamela Testa, aderente a Forza Nuova, dopo essersi evidenziata in occasione di manifestazioni no mask, e, infine, Biagio Passaro, tra i *leader* del movimento IoApro. Informo che sono in corso serrate attività di indagine e verifiche dei filmati registrati dal sistema di videosorveglianza per individuare altri responsabili di condotte penalmente rilevanti in relazione ai fatti accaduti presso la sede della CGIL. Tali attività hanno portato ieri sera all'esecuzione di misure di custodia cautelare in carcere nei confronti di ulteriori riconosciute grazie alle immagini che li ritraggono durante l'assalto alla sede sindacale. Si tratta di Massimiliano Ursino e Lorenzo Franceschi, appartenenti entrambi al sodalizio Forza Nuova, accusati di devastazione e saccheggio in concorso con altri e di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Un ulteriore punto da approfondire è poi rappresentato dall'inedito tentativo di portare effettivamente l'assedio a Palazzo Chigi e a Montecitorio, dando così seguito a propositi quasi di carattere insurrezionale, minacciati anche in precedenza attraverso i *social*. Per lunghe ore una fiumana di manifestanti, provenienti in prevalenza da Via del Tritone, ha tentato, a più riprese, di avvicinarsi alla Presidenza del Consiglio dei ministri con intenti palesemente ostili. Gli scontri si sono poi susseguiti nell'adiacente Via del Corso e anche in prossimità di Largo Goldoni, laddove i manifestanti hanno eretto improvvisate barricate al riparo delle quali hanno lanciato oggetti contundenti all'indirizzo delle Forze dell'ordine. Nell'occasione gli assalti, come hanno mostrato le immagini in diretta televisiva, sono stati contenuti con l'impiego di lacrimogeni, di mezzi speciali, idranti; si è dovuto ricorrere a cariche di alleggerimento per disperdere i manifestanti più esagitati allorché i loro tentativi di sfondamento si facevano più intensi e pericolosi. Tra le Forze di polizia si sono alla fine contati - come ho detto - 41 feriti, 11 dei quali appartenenti alla questura capitolina, 21 al reparto mobile di Roma, 3 all'Arma dei carabinieri, 6 alla Guardia di finanza. In occasione degli scontri si è proceduto all'arresto in flagranza di altre sei persone, cinque delle quali per violenza, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale e una per lesioni personali aggravate dall'uso di arma impropria. Il dispositivo di sicurezza che ha protetto le sedi istituzionali più rappresentative e quelle del Governo nazionale e del Parlamento ha, dunque, fronteggiato una situazione che, per dimensione, intensità e durata, non ha avuto precedenti. La giornata del 9 ottobre si è conclusa registrando presso il pronto soccorso del Policlinico di Roma un ulteriore episodio collegato ai disordini avvenuti nel pomeriggio. Intorno alle ore 24, alcuni familiari di Paolo Marchetti, manifestante rimasto contuso nei tafferugli e sottoposto a *triage* per le cure del caso, cercavano di raggiungere il loro parente, il quale, dopo aver riferito di non essere vaccinato, aveva anche rifiutato di sottoporsi al tampone. I parenti del Marchetti, inveendo all'indirizzo dei sanitari, tentavano anche un accesso forzoso all'interno del pronto soccorso, non riuscito grazie all'intervento degli agenti della Polizia di Stato, presenti occasionalmente sul posto per le necessarie cure mediche determinate dall'incidente avvenuto poco prima. In quel frangente, lo stesso manifestante dava in escandescenza, aggredendo il personale infermieristico e spintonando un operatore sanitario che tentava di fermarlo. Il Marchetti si è poi allontanato dall'ospedale unitamente ai suoi familiari; la Digos sta svolgendo un'attività di indagine per valutare gli aspetti penali delle condotte venute in rilievo durante l'episodio, che comunque non ha comportato la devastazione dei locali sanitari, come richiamato da alcune testate giornalistiche. Passo ora a riferire sui fatti accaduti sabato scorso a Milano. Nel primo pomeriggio, intorno alle ore 16, si è radunato a Piazza Fontana un folto numero di manifestanti che protestavano contro l'introduzione delle certificazioni verdi. La composizione dei partecipanti è risultata, come di solito, molto variegata, con la parte più consistente priva di una precisa connotazione e con la presenza di un gruppo di circa 80 persone riconducibili all'area anarchica. L'iniziativa ha visto l'immediato intervento delle Forze di polizia, le quali hanno provveduto a predisporre nuclei di sbarramento sulle principali vie di uscita dalla piazza, avvertendo i partecipanti che la stessa iniziativa avrebbe potuto proseguire solo in forma statica e delle conseguenze legali della inosservanza di tali indicazioni. La manifestazione, che ha visto l'iniziale partecipazione di qualche migliaio di persone, già intorno alle 17 raggiungeva le 3.000 unità. Poco dopo i manifestanti, interloquendo con i responsabili dell'ordine pubblico, hanno espresso l'intenzione di volersi indirizzare verso la camera del lavoro, ma è stato categoricamente escluso che tale destinazione potesse essere ricompresa in qualunque forma dinamica della protesta. Alle 17,30 i dimostranti si sono mossi in direzione di Piazza Duomo, ove nel frattempo si era provveduto a proteggere i punti più sensibili, proseguendo quindi per Piazza San Babila e lungo Corso Venezia, sino a giungere in Piazza Oberdan. In quel frangente, con ulteriori contingenti di forza pubblica, coordinati da funzionari, si è provveduto anche a proteggere la sede del quotidiano «Libero», già oggetto di contestazioni in precedenti analoghe manifestazioni. Vi è da dire che l'iniziativa, intanto, vedeva incrementare i partecipanti, raccogliendo in quel momento 8.000 unità circa. È in questa fase che uno sparuto gruppo di militanti anarchici ha tentato di proseguire verso Corso Buenos Aires. Tuttavia, tale improvvisa deviazione è stata fronteggiata e impedita, grazie all'invio di un ulteriore contingente di polizia, rimasto sul posto fino al completo passaggio dei manifestanti. Nello stesso momento, circa 80 anarchici, appartenenti al centro sociale Telos di Saronno, raggiungevano la testa del corteo, per tentare un'ulteriore deviazione verso la sede della Regione Lombardia. Anche in questo caso, però, venivano prontamente bloccati, mentre intanto si provvedeva a proteggere quella sede istituzionale con un apposito presidio. Anche successivamente, i manifestanti, con ripetuti tentativi di deviazione del corteo, hanno provato a indirizzarsi verso altri obiettivi, tra i quali la sede del «Corriere della Sera», la camera del lavoro, il tribunale e Assolombarda. Anche queste continue e ripetute manovre, che intendevano trascinare le Forze di polizia verso uno scenario di guerriglia urbana, sono state contenute e respinte, in virtù di un notevole dispendio di energie necessario a proteggere tutti i vari possibili obiettivi, tra i quali anche quello della Stazione Centrale, opportunamente presidiata. I fatti accaduti a Milano, durati diverse ore, hanno creato una prolungata situazione di disagio alla cittadinanza sia per il blocco veicolare, che in taluni momenti ha compromesso la circolazione, sia per il clima di tensione che ha interessato le principali vie del centro. In occasione della manifestazione sono stati eseguiti due arresti in flagranza per resistenza aggravata a pubblico ufficiale, per i quali è già avvenuta la convalida, nonché fermi per identificazione per altrettanti soggetti indagati per i reati di violenza privata, interruzione di pubblico servizio e mancato preavviso di manifestazione. Informo che eventuali responsabilità verranno accertate anche con riferimento a ulteriori 66 persone, la cui posizione è attualmente al vaglio dell'autorità giudiziaria. a quanto è avvenuto ieri mattina a Trieste, ritengo sia necessario un preliminare chiarimento. La manifestazione era stata preceduta da un'intensa attività di confronto e di mediazione che ha visto impegnati, per diversi giorni, il prefetto di Trieste, il presidente della locale autorità portuale in uno strenuo tentativo di scongiurare che l'iniziativa di blocco delle attività dello scalo giuliano venisse attuata e ciò in considerazione dei gravi danni che ne avrebbe sofferto non solo quell'importante sito della logistica, ma anche l'intera filiera produttiva e distributiva che vi è collegata. L'iniziativa era stata assunta dal coordinamento lavoratori portuali Trieste che ha, peraltro, una rappresentanza dei lavoratori minoritaria ed è stata immediatamente oggetto di strumentali adesioni da parte di ambienti ideologizzati, in particolare della sinistra antagonista, sebbene non sia mancata una marginale presenza della destra radicale. Elemento, quest'ultimo, che fa riflettere rispetto a quella trasversalità politico-ideologica della protesta no *green pass*, capace di far convergere formazioni e gruppi anche contrapposti sull'obiettivo comune della violenta opposizione alle istituzioni e alle misure di prevenzione sanitaria. Tengo anche a precisare che la proclamazione dello sciopero indetto per ben cinque giorni, cioè dal 15 al 20 ottobre, era stata oggetto di una comunicazione da parte della commissione di garanzia per l'attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, che ne aveva rilevato l'illegittimità, sia sotto il profilo del mancato rispetto del termine del preavviso sia sotto quello dell'inosservanza della regola della rarefazione oggettiva, preordinata a evitare gravi pregiudizi alla continuità del servizio e relativi riflessi sull'utenza. Nonostante il richiamo del prefetto di Trieste alla palese illegittimità dello sciopero e ai risvolti di illiceità che vi erano connessi, dal 15 ottobre è stato attuato un presidio al varco 4 del molo VII del Porto di Giuliano, che ha visto nella sua punta massima la presenza di 8.000 manifestanti. Grazie, tuttavia, all'utilizzo degli altri varchi disponibili, le attività portuali cui ha potuto accedere la stragrande maggioranza dei lavoratori in disaccordo con la protesta - non hanno subito un blocco e hanno continuato a svolgersi regolarmente, seppure registrando alcune criticità. La presenza a Trieste - divenuta polo di attrazione della protesta contro il *green pass -* di migliaia di manifestanti, provenienti anche da altre Regioni d'Italia, è proseguita anche nelle giornate di sabato 16 16 e domenica 17, di fatto impedendo a oltre 700 mezzi pesanti di raggiungere l'area portuale per effettuare le operazioni di carico e scarico, nonché di eseguire lo sbarco delle merci da una nave attraccata allo stesso molo VII. A fronte di tale situazione, nel pomeriggio di domenica 17 ottobre, il prefetto di Trieste ha indetto un comitato urgente per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza dei vertici locali della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e dell'autorità portuale nonché del procuratore della Repubblica. Si è condiviso in quella sede di effettuare per la mattina seguente lo sgombero del varco 4, in considerazione dei disagi già accusati e destinati ad aggravarsi. Alle 8,30 di lunedì 18, pertanto, hanno avuto inizio le operazioni di sgombero dell'area portuale interessata e, nonostante il ripetuto invito del dirigente del servizio di ordine pubblico a liberare il sito, i manifestanti hanno improvvisato un *sit-in*, bloccando l'avanzamento di uomini e mezzi e hanno anche rifiutato la proposta di trasferirsi in un'altra piazza per continuare in quella sede la protesta. Nei momenti di maggiore tensione, in cui si è prefigurato il chiaro pericolo di una degenerazione della situazione dell'ordine pubblico, è stato necessario ricorrere all'uso dei mezzi idranti e dei lacrimogeni, per superare la resistenza opposta dai manifestanti più esagitati. Si è fatto ricorso a un intervento tecnico-operativo, che ha avuto caratteristiche analoghe a quelle già illustrate in relazione ai fatti di Roma, accaduti in prossimità di Palazzo Chigi e Montecitorio. Anche durante le fasi più concitate, il confronto con i manifestanti è stato sostenuto con moderazione e modalità di contenimento della forza, come dimostra il fatto che nonostante la presenza di migliaia di persone, la gran parte del tutto estranea alle maestranze portuali, non si siano registrati che pochissimi casi di malore - tre soltanto - tra i partecipanti dovuti allo stato di panico per la rissa. Tre operatori del reparto mobile hanno riportato lievi contusioni. A seguito dello sgombero dell'area portuale, la protesta, con la presenza di circa 200 manifestanti, ha impegnato anche le zone attigue al porto e il centro cittadino in cui, per alcune ore del pomeriggio, si sono registrati tafferugli con le Forze di polizia al cui indirizzo sono stati lanciati sassi e bottiglie. Allo stato risultano deferite all'autorità giudiziaria quattro persone per i reati di interruzione di pubblico servizio e istigazione a disobbedire alle leggi, nonché per mancato preannuncio di manifestazione. Sono in corso attività di indagine per identificare eventuali altri autori di condotte delittuose. Nella serata di ieri una delegazione del comitato di coordinamento lavoratori portuali di Trieste insieme ad altri rappresentanti del variegato mondo dei *no green pass* sono stati ricevuti dal prefetto. In quell'occasione è stato chiesto di poter avere un incontro con un esponente del Governo a fronte dell'impegno a non riproporre il blocco delle attività portuali, a liberare Piazza Unità d'Italia, dove nel frattempo era stato istituito un presidio, e a spostarsi in un'area del porto vecchio. Dopo breve tempo è stata comunicata la disponibilità del ministro Patuanelli, sorretta ovviamente dal mantenimento degli impegni assunti. Informo che attualmente l'area portuale di Trieste è ritornata pienamente agibile e che non si registra alcuna criticità nelle attività dello scalo. La difesa dell'ordine pubblico ha sempre corrisposto a un impegno severo quanto delicato. Lo è divenuto in modo particolare in questo difficile periodo, in cui la protesta ha finito per investire minacciosamente pressoché ogni ambito: quello politico e sindacale come quello sanitario e scolastico, facendo emergere nuovi soggetti da tutelare e nuovi obiettivi sensibili da proteggere. Rileva anche il carattere sfidante di questa protesta, intenzionata a non fermarsi nonostante gli inviti alla moderazione e a proseguire a oltranza per raggiungere il suo scopo, organizzando presidi, fiaccolate e *sit-in*. L'obiettivo che dobbiamo prefiggerci è guidare il Paese ad uscire dalla pandemia, senza che le effervescenze della conflittualità producano traumi o ferite profonde. L'andamento delle manifestazioni svoltesi nell'ultimo fine settimana fa sì che non si possa in alcun modo abbassare la guardia e anzi induce a mantenere costantemente massima l'attenzione, per garantire che non sia turbata la tranquillità della comunità nazionale. Lo strumento per raggiungere questo obiettivo è garantire il doveroso equilibrio tra il diritto di manifestare anche il proprio dissenso e la tutela dei diritti di libertà dei cittadini, nel rigoroso rispetto dei principi costituzionali. Garantisco, nella mia responsabilità di Ministro dell'interno, in coerenza con i valori che hanno accompagnato la mia lunga esperienza al servizio della Repubblica, che tutti i cittadini potranno essere certi che questi due diritti saranno sempre tutelati nel rispetto dei principi democratici che sono alla base del nostro Paese.

Signor Ministro, le sue argomentazioni non sono state affatto convincenti. Dopo aver patrocinato pomposamente una manifestazione che si dichiarava antifascista, il Governo è andato a Trieste in una veste completamente opposta. Gli idranti e i lacrimogeni che hanno colpito i manifestanti pacifici hanno confermato la nascita di un nuovo regime. Lei, signor Ministro, volendo evitare disordini a Roma, ha scelto di non sbarrare la strada a Forza Nuova nel momento in cui ciò era indispensabile, dicendo di temere conseguenze sull'ordine pubblico, ma, sia a Roma che a Trieste, la polizia è intervenuta senza esitare con cariche e lacrimogeni su una folla di manifestanti miti. Dunque, se da una parte non si è mosso un dito per evitare a Piazza del Popolo le infiltrazioni fasciste che avevano preannunciato la devastazione della sede della CGIL, a Trieste abbiamo assistito a scene degne di un regime autoritario, con la polizia in tenuta antisommossa che punta gli idranti e lancia lacrimogeni contro cittadini inermi, che rivendicavano solo il diritto di manifestare. Evidentemente le infiltrazioni della destra eversiva non ostacolate erano funzionali allo screditamento di tutta la piazza e dell'intera posizione dei manifestanti no *green pass*, ma il popolo non è caduto nel tranello ed è tornato subito nelle strade per far sentire pacificamente la propria voce. Eppure a Trieste non si è esitato un attimo a sciogliere brutalmente un presidio di lavoratori che non chiedeva altro, se non la revoca di un provvedimento discriminatorio, che limita i diritti fondamentali, rischiando ritorsioni e sanzioni. Degli eventi di Trieste non mi meraviglia il silenzio complice di quei partiti ligi al neoliberismo senz'anima, che non ama il popolo, il rispetto dei diritti costituzionali e dei lavoratori, di cui Draghi è esponente di prima punta. Ciò che mi rattrista più di tutto è la convivenza di chi si professava diverso e diceva di voler restituire diritti alle fasce deboli e indifese della popolazione, arginando l'azione di poteri forti e *lobby* economico-finanziarie. Temo seriamente che in questo Paese si sia ormai consolidata la prassi di nascondere politiche a diretto vantaggio di una ristretta classe sociale dietro il manto dell'identità. In questo contesto è l'intero sistema democratico a essere sotto attacco. Lo svilimento del ruolo del Parlamento, organo di mera ratifica delle scelte del Governo, e la gestione delle manifestazioni a Roma e a Trieste rappresentano solo tristi, ma eclatanti esempi. C'è una sola strada percorribile per lei, signor Ministro, dopo i fatti di Roma e Trieste: le dimissioni. La posta in gioco in questo momento storico è altissima: siamo chiamati a decidere quale modello sociale vogliamo per noi e per i nostri figli nel prossimo futuro e quindi dobbiamo scegliere da che parte stare e resistere ancora contro ogni sopruso in forme pacifiche e non violente.

il Gruppo Forza Italia ovviamente coglie questa occasione per condannare i fatti gravissimi che si sono verificati sabato 9 ottobre a Roma, l'aggressione e l'occupazione alla sede della CGIL, le iniziative e le violenze

Abbiamo sentito la sua ricostruzione, signor Ministro, e mi meraviglia, come ho avuto modo di segnalarle più volte anche in via informale, l'impunità di cui hanno goduto alcuni soggetti, soprattutto sulla piazza romana. I protagonisti che lei ha citato più volte erano stati oggetto di segnalazione delle autorità di polizia e di alcuni settori della magistratura, mentre altri settori competenti non avevano Addirittura il protagonista, che lei ha citato, anni fa fu sorpreso con un quantitativo ingente di cocaina, una quantità rilevante che fu considerata a uso personale, benché fosse una quantità Quindi io mi chiedo perché questa sottovalutazione e questa impunità di alcuni gruppi e di alcune realtà. *(Applausi)*. Questo attiene anche alla magistratura romana, va detto; impunità che anche altri settori della sinistra hanno avuto. Noi non abbiamo dubbi sulla matrice di quello che è successo a Roma e sulla responsabilità prevalente di gruppi neofascisti e di estrema destra, che hanno trovato l'occasione di una platea vasta, che non era ovviamente tutta composta da loro aderenti (non ne hanno così numerosi) e che hanno potuto in qualche modo orientare, esagitare e strumentalizzare. Io credo, signor Ministro, che sia giusto vedere a 360 gradi; è quello che il Gruppo Forza Italia ha detto in questi giorni e che penso dirà anche domani. Lei ha citato i 41 poliziotti feriti dagli estremisti a Roma. Io voglio ricordare insieme a loro - e ringraziare quegli appartenenti alle Forze dell'ordine - le centinaia di carabinieri e poliziotti feriti in Val di Susa in questi anni. *(Applausi)*. C'è uno stillicidio settimanale, di fronte di fronte al quale non vedo invocare scioglimenti, che poi le autorità competenti decideranno se essere attuati o attuabili; noi non abbiamo velo rispetto a questo e non dobbiamo difendere chicchessia. Un po' di sottovalutazione - diciamo così - c'è stata e la ringrazio per una ricostruzione onesta, perché capisco le difficoltà del suo ufficio. Fare il Ministro dell'interno è un compito gravoso e lei che ha ricoperto tanti incarichi credo che lo abbia in questi mesi constatato. Però indubbiamente invito il Governo a non sottovalutare nessuna situazione.

della legalità e della lotta all'impunità. *(Applausi)*. Lo dico anche per i fatti di Trieste. Non ho capito ancora la strumentalizzazione a Trieste, da parte di alcuni portuali, della vicenda del *green pass* e quant'altro. Non c'entrava niente; non era una lotta sindacale di lavoratori per il loro posto di lavoro, che avremmo rispettato. *(Applausi)*. un po' maniacale, sinceramente. Per carità, ognuno può fare quello che vuole; però poi c'è la legge e quindi credo che l'intervento sia stato necessario. Noi invitiamo il Governo a non sottovalutare nulla. Inviterei il signor Ministro e anche il Presidente del Consiglio ad accettare una proposta che Forza Italia fa da tempo: un incontro di maggioranza con i Ministri competenti sui temi dell'ordine pubblico e dell'immigrazione. *(Applausi)*. Noi apprezziamo il Presidente del Consiglio, ma ci metta un po' di faccia sui temi dell'immigrazione e della sicurezza. È un Governo nato per vaccinare e per fare i piani per l'Europa; però anche queste sono questioni. Voglio infine dire, signor Ministro, che noi presenteremo delle proposte per una maggiore tutela delle Forze di polizia, che non possono essere aggredite. *(Applausi)*. Oggi durante una manifestazione - ho finito, signor con un telefonino si riprende il poliziotto che reagisce, forse eccessivamente. Ma non hanno fatto vedere che a quel poliziotto, cari colleghi, avevano spaccato il naso pochi minuti prima. Le immagini vanno mostrate tutte, anche quelle delle aggressioni ai carabinieri e ai poliziotti. Poi, se le reazioni sono improprie, saranno sanzionate; ma non è che si possono usare, durante le manifestazioni, strumenti da parte di giornalisti o manifestanti per mostrare alcune cose e altre no. È necessario più controllo anche sui *social*, signor Ministro. Forse bisogna modernizzare qualche apparato; gli strumenti tecnici ci sono e nessuno va censurato, ma chi usa mezzi di progresso e di comunicazione per fomentare la violenza...

Signora Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, signora Ministra, vorrei iniziare questo mio intervento dichiarando la solidarietà mia e del Gruppo al quale appartengo, il MoVimento 5 Stelle, alle Forze dell'ordine, che hanno subito attacchi e feriti (se ne ricordava prima il numero). Noi siamo assolutamente dalla parte delle Forze dell'ordine. *(Applausi)*. Nel contempo, voglio esprimere solidarietà a tutti quei manifestanti pacifici che hanno esercitato un loro diritto costituzionalmente garantito. Noi siamo in una Repubblica democratica e quindi chiunque deve poter dimostrare e portare avanti la propria voce, anche se nello specifico possiamo non

epoche terribili e buie, in cui si assaltavano le camere del lavoro e i sindacati e si attaccavano i lavoratori. A quei periodi e a quelle epoche non vogliamo più tornare e quindi dobbiamo stare attenti e analizzare ciò che sta succedendo in questo momento. Quello alla sede della CGIL è un attacco di chiara matrice fascista e non lo dico io, ma gli stessi elementi che hanno portato a compimento quel vile attacco, che si dichiarano apertamente fascisti. A volte si definiscono fascisti del terzo millennio o semplicemente fascisti: lo dicono loro. Ebbene, non dovremmo consentire consentire che ci sia questa voglia di nuovo squadrismo e questa voglia di imporre le proprie idee con la violenza. Se si vogliono propalare le proprie idee, si può farlo rispettando i limiti e i principi della nostra Costituzione, giammai utilizzando la violenza. Peraltro devo anche sottolineare che, nei mesi scorsi, una parte consistente della destra, presente anche in Parlamento, a mio giudizio ha soffiato sul fuoco. Ricordo le parole che sono state ripetute migliaia di volte, in cui si gridava alla dittatura sanitaria e in cui le mascherine che tutti portiamo ancora oggi venivano definite museruole. Quello, dal mio punto di vista, è stato un atteggiamento fortemente sbagliato, che ha avuto un'evidente ricaduta su alcuni gruppuscoli, che non cercano

cui partecipavano 20 o 30 persone. È chiaro che aver soffiato sul fuoco in quel modo per tanto tempo ha portato alla situazione odierna. se si vuole essere una forza politica responsabile, che obbedisce alle nostre regole democratiche, non si può un giorno indossare la felpa della Polizia e il giorno dopo

gridavano alla strategia della tensione e alla voglia di mettere il Paese in una determinata situazione.

però dirci, sempre per essere chiari con noi stessi, che nell'assalto alla CGIL si sono evidenziate delle falle molto gravi nel sistema di sicurezza e quindi, specialmente in specialmente in vista di importanti appuntamenti internazionali per il nostro Paese, come per esempio quello del G20, è assolutamente necessario tutelare il diritto a manifestare pacificamente, per prevenire ogni forma di violenza, sia quella fascista, sia quella di qualsiasi altra origine. Concludendo, signor Presidente, il MoVimento 5 Stelle chiede di calmierare immediatamente il prezzo dei tamponi e di valutare, nel giro di qualche settimana, la proporzionalità delle misure adottate, alla luce della nuova situazione epidemiologica e del *trend* di vaccinazione. Riteniamo queste valutazioni assolutamente essenziali, proprio per ridare tranquillità al Paese e tener conto di come stanno andando la pandemia e le misure di contrasto messe

Signor Presidente, colleghi, Ministro, ho chiesto di intervenire *in extremis* perché alcune sue parole mi hanno veramente ferito. Lei è riuscita con pochi passaggi del suo discorso a offendere *in primis* le Forze di polizia che lei rappresenta,

È un poliziotto che si rende credibile agli occhi dei manifestanti. Non è credibile cinque minuti dopo mentre picchia in maniera inconsueta un ragazzo a terra già immobilizzato. Dovrebbe quindi spiegarci le ragioni della seconda fase dell'azione di quel poliziotto. detto benissimo, è stata monopolizzata da 200 criminali che non hanno nulla a che vedere con nessuna forza politica e nessuna azione politica. Penso che il fascismo, anche il più estremo, non abbia niente a che fare con un invasato cocainomane che dovrebbe stare

onorevoli colleghe e colleghi, desidero ringraziare anzitutto la Ministra per la sua presenza in quest'Aula perché è estremamente importante dare il giusto peso agli episodi che sono accaduti.

quando si fanno le riprese bisognerebbe sempre riprendere tutto l'episodio e il contesto nel quale le vicende accadono e non inquadrare invece la reazione di un singolo poliziotto che magari è stato sottoposto ad azioni di violenza poco prima assieme ai suoi colleghi. Questo è necessario dirlo a difesa dell'operato delle Forze dell'ordine che, quotidianamente, a difesa delle istituzioni, mettono a repentaglio la loro vita loro vita per tutti quanti noi, per la popolazione e la difesa dei valori democratici che noi siamo obbligati doverosamente a tutelare. I fatti dello scorso ottobre, come lei ha ricordato con una relazione estremamente esaustiva, sono stati connotati da una violenza e da una gravità inaudita. Quella che avrebbe dovuto essere una manifestazione pacifica contro l'obbligo del *green* *pass* per i lavoratori si è trasformata in un vero e proprio attacco squadrista a causa della presenza di soggetti appartenenti a Forza Nuova ed altre organizzazioni notoriamente di estrema destra. Prima gli scontri con la polizia, poi i numerosi episodi di violenza che sono culminati con il danneggiamento della sede della CGIL di cui ho parlato, ed anche con le aggressioni al personale sanitario del Policlinico, dove era stato condotto uno dei partecipanti alla protesta in stato di fermo. Di questi fatti mi hanno colpito soprattutto due elementi. Il primo

al lavoro e ad un'istituzione che tutela i lavoratori. La democrazia e la tutela dei lavoratori non sono però cosa da poco, da affrontare a cuor leggero. Lo testimonia, credo in maniera inequivocabile, la manifestazione pacifica che si è svolta sabato scorso e che ha visto protagonisti - per l'appunto - moltissimi lavoratori, le principali sigle sindacali, moltissimi partiti politici - come dicevo - i lavoratori che attorno al concetto di democrazia si sono ancora una volta stretti assieme a tutti noi. Abbiamo partecipato convintamente a quelle manifestazioni e c'eravamo proprio perché gesti come quelli accaduti il 9 ottobre si pongono in netto contrasto con lo spirito democratico che guida il nostro Paese.

Le parole che sono state dette "portateci da Landini o lo andiamo a prendere noi" sono di una gravità inaudita e dovrebbero davvero farci riflettere su qual è l'ideologia e su quali sono le intenzioni di queste persone.

Senza timore di essere smentito, mi permetto di affermare che questi episodi sono da inquadrare nel canone dello squadrismo armato, di cui si avvalse il fascismo (purtroppo ne abbiamo tristi ricordi)

che va ad incidere in un particolare momento storico nel cuore delle istituzioni democratiche di questo Paese. Non posso non pensare che questi episodi si sono verificati nel momento in cui il Paese ha dato segnali di ripartenza. Non posso non pensare che non sia voluto questo attacco al cuore delle istituzioni, soprattutto a una delle principali

Speravo ci fosse una condanna unanime delle violenze che ci sono state, così invece non è stato. Mi dispiace dover rimarcare una cosa: io non sono solito criticare in maniera gratuita le affermazioni dei colleghi, perché ho rispetto estremo delle idee di ciascuno, ma francamente mi lasciano molto perplesso e voglio pensare siano il frutto di una scarsa informazione, considerata anche la giovane età. Chi come me ha ormai i capelli bianchi sa cosa vuol dire parlare di strategia della tensione e sa cosa ha voluto dire nel nostro Paese affrontare quel periodo della strategia della tensione. Infatti, riportare alla memoria in maniera del tutto incauta e inappropriata quella terminologia e quel periodo

con la difesa a costo della propria vita. Come dicevo - e lo ribadisco - le Forze dell'ordine, qualunque esse siano, quotidianamente mettono a repentaglio la propria vita nel nostro interesse, nell'interesse dell'intera cittadinanza. Tuttavia è evidente che chi parla a vanvera - mi si passi il termine forse poco cortese poco cortese - di strategia della tensione non sa di che cosa parla e ho idea che si lanci in affermazioni di questo genere soltanto soltanto per cercare di coprire quel che è effettivamente accaduto il 9 ottobre. Di fronte a questi fatti la nostra condanna è netta.

persone. I fatti del 9 ottobre vanno condannati. Sui profili penali della vicenda deciderà la magistratura come è corretto che sia, ma è arrivato il momento, qui dentro, di decidere cosa vogliamo fare di queste persone che stanno veramente minando o tentando di minare il nostro sistema democratico. Personalmente, sono convinto che ci riusciremo ancora una volta, perché credo che la coscienza democratica che abbiamo maturato, soprattutto dopo gli anni di piombo,

Ministro Lamorgese, oggi dobbiamo accertare che purtroppo la patologia da cui è affetta questa meravigliosa Nazione

che lei fa vedere ogni giorno. Da una parte ha mostrato una faccia quando non è riuscita a fermare un *rave* illegale fatto su un terreno privato

senza il quale - lei sa benissimo - non si possono accompagnare i bambini a scuola, non si può bere il caffè al bar. Quella faccia, signor Ministro, che in una Nazione così lacerata e sofferente ha lasciato che migliaia di ragazzi italiani e stranieri si riunissero in un *rave* illegale, in quel caso davvero senza alcun tipo di sicurezza, usando qualsiasi tipo di droga in commercio.

Non si spiegherebbero altrimenti le due facce del suo Ministero. Perché accanto al *rave* e alle chiusure per Covid, invece una cosa certa...*(Commenti).* Va bene, ma non è importante. Per cortesia, non c'è bisogno di fare polemica. Faccia continuare la senatrice Garnero

del problema delle periferie. È stato rotto il patto sociale con i cittadini che si sentono abbandonati, anche perché voi accogliete - o, meglio, abbandonate - gli immigrati nelle periferie. Questa è la ragione della paura degli italiani. Poi, naturalmente, c'è la faccia del Ministero, che lei ha molto ben rappresentato nell'Aula della Camera quando ha risposto ai quesiti di Giorgia Meloni in merito all'aggressione alla sede della CGIL, cui - lo ribadisco - va tutta la nostra solidarietà.

Lei sapeva anche che il rischio di degenerazione in atti di violenza era altissimo. Lei, signor Ministro, ha quindi scelto di lasciare sette poliziotti a prendere le botte davanti alla CGIL. Lei, Ministro, ha scelto di non proteggere la sede del sindacato. Lei, signor Ministro, ha scelto di non tutelare chi ha il sacrosanto diritto di manifestare in maniera pacifica pacifica per la propria libertà. Le vorremmo chiedere a chi faceva comodo quell'incidente. A quale propaganda?

ha un'altra faccia e, quindi, nel porto di Trieste, anche se non vi è stato alcun tipo di incidente, non si poteva e non si può manifestare.

Il Ministero cosa fa? Manda gli idranti e i lacrimogeni. Chiedo ai colleghi: se fossimo stati noi a mandare gli idranti e i lacrimogeni, che cosa sarebbe successo? Purtroppo, o per fortuna quella cultura a noi non appartiene; a voi appartiene la cultura degli idranti e dei lacrimogeni. *(Applausi)*. Allora, qui il pugno duro sì, altrove no. I ragazzi del *rave* le facevano più o meno paura, signor Ministro? Ci faccia capire. Siamo una Nazione in cui, ogni tre venerdì, c'è uno sciopero degli aerei e dei trasporti perché la protesta e gli scioperi sono un diritto. Oppure è cambiato qualcosa e non sono più un diritto lo sciopero, né la protesta? Ci può spiegare quali sono le regole? infatti la protesta violenta su cui chiudete gli occhi finché non degenera (anzi, andate anche oltre) e poi c'è l'altra protesta, pacifica, che va fermata con i lacrimogeni. Ma voi vi dovete vergognare di come state riducendo questa Nazione! Lo sciopero è legittimo

abbiamo un po' di confusione. Questo è un Governo che mischia tutto, chiacchiera di sostegno agli anziani e poi taglia le pensioni. È una maggioranza che certifica con i numeri il fallimento del reddito di cittadinanza, ma poi non lo abolisce; una maggioranza - diciamoci la verità - che vorrebbe arrivare all'obbligo vaccinale, ma poi non ha il coraggio politico per imporlo. Questo state facendo: vi state nascondendo dietro il *green pass*,

Andate forse a sgridare gli scolaretti che buttano per terra la carta davanti alle scuole e magari date una pacca agli spacciatori? Che faccia ci mostra oggi, ministro Lamorgese? Sia chiara una volta per tutte, con parole di verità.

puntuale ed esauriente. D'altra parte, i suoi detrattori hanno dovuto parlare di *rave*, di immigrati, di Linus e di altre amenità, perché difficilmente è possibile smentire le cose che ha detto. Voglio partire da un dato, che è stato citato anche da lei nella sua relazione: dall'inizio della pandemia, nel nostro Paese si sono svolte oltre 5.700 manifestazioni di piazza, di cui 3.700 solo quest'anno. Quasi tutte si sono svolte senza problemi, garantendo la possibilità e il diritto di manifestare a tutti, senza che questo comportasse violenze o danneggiamenti. Se confrontiamo questi dati con ciò che è avvenuto in molti altri Paesi, a partire per esempio dalla Francia dove la gestione delle piazze è stata molto più complicata e gli incidenti molto più frequenti,

che con equilibrio hanno saputo gestire al meglio situazioni spesso difficili. Non lo dico per non affrontare o minimizzare ciò che è successo o per nascondere l'assalto alla CGIL o i recentissimi episodi di Trieste e di Milano. Lo ricordo perché, a fronte di una capacità generalizzata

i fatti di Roma per attaccare quotidianamente un'autorità dello Stato, la ministra dell'interno Lamorgese. Si getta discredito su apparati pubblici che per due anni hanno operato bene, con equilibrio, per difendere i cittadini e garantire il diritto di manifestare in un clima sempre più di coesione, sempre più di E lo si fa rischiando di confondere le responsabilità dei violenti e quelle delle Forze dell'ordine. Gli attacchi continui al Ministro sono talmente strumentali che mi domando se non servano a evitare di fare i conti con ciò che tutti dobbiamo fare: prendere le distanze concretamente e senza ambiguità dai violenti, tutti i violenti. La narrazione che, sempre per attaccare la Ministra, si è cercato di imporre e che racconta che è il Ministro dell'interno a decidere i movimenti e le scelte delle Forze dell'ordine in piazza, a comandare la piazza, è palesemente falsa; l'ho sentita raccontare anche adesso. Ricordo solo un precedente drammatico di un Ministro che ha seguito dalla centrale operativa della questura una manifestazione: era il G8 di Genova. Per il resto, tutti noi sappiamo che quella di Roma era una manifestazione non autorizzata che la responsabilità delle scelte che vengono fatte per garantire lo svolgimento delle manifestazioni è di chi comanda le Forze dell'ordine in piazza ed è in grado di valutare meglio di chiunque altro la situazione. Oggi il Ministro ha ribadito le ragioni che hanno portato i responsabili della catena di comando a fare le scelte - alcune delle quali discutibili che sono state fatte a Roma e che hanno portato anche - lo dobbiamo dire - a difendere Palazzo Chigi, a difendere le istituzioni, ma anche ad esporre in misura eccessiva, inaccettabile, la sede della CGIL, fino a consentire l'inaccettabile invasione della stessa. La solidarietà al sindacato da questo punto di vista non basta. Al Ministro vogliamo chiedere di andare avanti e fare chiarezza su quanto successo, sulle responsabilità responsabilità e sugli errori, se ce ne sono stati, perché questo ci serve per non ripeterli, sapendo che la fase difficile, la fase di tensione in questo Paese probabilmente non è finita. Se errori ci sono stati, vanno sottolineati e ancora di più, signora Ministra, serve per capire perché non si è potuto prevedere e prevenire ciò che è successo. Noi vogliamo chiarezza sui fatti, come lei - ci ha spiegato - sta cercando di fare, ma dire che siamo di fronte a una volontà del Governo di provocare incidenti per alimentare tensioni è grave, inaccettabile e indimostrabile. *(Applausi)*. Ancora una volta, facendo così, Ancora una volta, facendo così, in nome della propaganda, si mette in discussione la credibilità delle istituzioni, che in questo momento è fondamentale. Si offendono le Forze dell'ordine, perché non si sta con loro. Non si esprime solidarietà alle Forze dell'ordine se poi si pensa che siano parte di un disegno che vuole alimentare tensioni. Le tensioni di questi giorni vanno affrontate, confrontandosi con le ragioni di chi protesta, ma isolando e perseguendo i violenti. Sono loro, le organizzazioni neofasciste che hanno infiltrato e utilizzato la piazza di Roma, il nemico da battere. C'è chi vuole approfittare della rabbia o del disorientamento di alcuni per colpire le istituzioni; sono costoro i nemici, non certo la ministra Lamorgese, che continua a lavorare nell'interesse del Paese. Su questo non possono esserci non possono esserci ambiguità, timidezze o benaltrismi vari e non bisogna abbassare la guardia; anzi, dalle Camere oggi deve uscire un messaggio chiaro agli operatori delle Forze dell'ordine, che si sacrificano ogni giorno per garantire il diritto di manifestare in sicurezza, pacificamente. Dobbiamo dare il messaggio che tutte le istituzioni sono al loro fianco, a fianco dei manifestanti pacifici, a fianco delle Forze dell'ordine. E un messaggio chiaro deve arrivare anche a chi vuol fare delle legittime proteste un'occasione di violenza: le istituzioni sono più forti di loro e sapranno restare unite per contrastare con determinazione ed equilibrio tutti violenti.

signor Ministro, colleghe e colleghi, intanto voglio ringraziare il Ministro per la sua corposa ed esaustiva

del 9 ottobre a Roma. Sono passati ormai dieci giorni da quel 9 ottobre, ma quella data resterà impressa nella nostra storia. Era già accaduto cento anni fa che squadracce fasciste assediassero e devastassero le camere del lavoro. Allora lo Stato non si oppose e ci fu la marcia su Roma e il regime fascista. Addirittura, Gaetano Salvemini, come è stato ricordato, solo con l'omicidio Matteotti si rese conto di quanto per anni avesse sottovalutato quel tremendo pericolo per la democrazia. Oggi la reazione c'è stata, con gli arresti, ma anche con la straordinaria risposta popolare di sabato scorso a Roma promossa dai sindacati. Bene ha fatto il presidente Mattarella a evidenziare la fortissima reazione del Paese all'assalto alla sede del sindacato. So bene che all'ordine del giorno di oggi non c'è la richiesta dello scioglimento delle organizzazioni fasciste, che discuteremo domani, ma proprio lei, nella sua ricostruzione del sabato fascista, ci fornisce gli elementi per sostenere la nostra richiesta, forti della disposizione transitoria della Costituzione italiana. Dunque, vengo alla sua informativa. Sono più che legittimi gli interrogativi sul 9 ottobre. Appare chiaro, innanzitutto, che qualcosa non ha funzionato nella gestione dell'ordine pubblico. C'è stata sottovalutazione e, di conseguenza, inadeguatezza da parte delle Forze dell'ordine nel fronteggiare proprio quelli che lei, a caldo, ha definito segnali eversivi. Proprio lei ha fornito, poco fa, i numeri di quel 9 ottobre. Non vi aspettavate una partecipazione così numerosa alla manifestazione, perché le altre manifestazioni di no *green pass* e no vax dei sabati precedenti non erano state così consistenti. Vi aspettavate 3.000-4.000 persone: ne sono arrivate il triplo e, quindi, gli 840 uomini e donne delle Forze dell'ordine erano insufficienti. Piazza del Popolo questa volta era piena. Piazza del Popolo è stato un errore: troppo vicina ai palazzi delle istituzioni. Un anno fa, prima del *green pass*, in piena pandemia e *lockdown*, Roberto Fiore, *leader* di Forza Nuova, oggi in carcere, alla vigilia della manifestazione di Napoli, il 24 ottobre del 2020 scriveva in un *tweet*: «Che si accenda a Napoli la prima scintilla di rivoluzione contro la dittatura sanitaria». Quella stessa notte Forza Nuova pubblicò le foto della guerriglia cittadina: «Noi in strada a Roma; da Napoli partita la rivolta». Certo, è vero ed indubitabile che abbiamo garantito la libertà di manifestare. Lei ha citato 5.700 manifestazioni, ma in questi mesi vanno ricordati anche degli altri episodi violenti avvenuti nei cortei no vax Per brevità ne cito uno: il 28 agosto, a Roma, due manifestazioni, la prima a Piazza del Popolo e l'altra alla Bocca della Verità. A Piazza del Popolo, più di duecento militanti di Forza Nuova tentano di superare lo sbarramento delle Forze dell'ordine, con cariche di alleggerimento per disperdere i neofascisti. Senza dimenticare il *gazebo* distrutto a Milano del MoVimento E voglio ricordare anche i numerosi giornalisti, cui va la nostra solidarietà, picchiati e insultati in queste manifestazioni. Signor Ministro, queste di estrema destra sono frange, lo sappiamo, non rappresentano l'intero movimento no *green pass*. Commetteremmo un errore a pensare che queste piazze non vadano ascoltate, perché esprimono un disagio sociale con il quale bisogna fare i conti. Non possiamo, però, non sottolineare la gravità della situazione, con le minacce a personalità politiche e del mondo scientifico impegnate nella battaglia contro la pandemia. Campagne di odio sui *social media*, pedinamenti fisici e minacce, come capitato all'infettivologo Matteo Bassetti, primario del San Martino di Genova. Questi distinguo, anche all'interno della maggioranza, questo cavalcare la protesta da parte della destra, sono pericolosi. Non c'è da contrastare nessuna dittatura sanitaria; non c'è nessuna libertà calpestata. Quanto successo il 9 ottobre a Roma segna un punto di non ritorno. In Corso d'Italia non c'era il popolo disorientato, impaurito dalla pandemia. Il 9 ottobre, sul palco di Piazza del Popolo, c'era il sorvegliato speciale Giuliano Castellino. Il 9 ottobre c'erano Roberto Fiore e Luigi Aronica, tra i fondatori dei NAR di Fioravanti e Mambro. Lo abbiamo ascoltato tutti Giuliano Castellino arringare la folla e annunciare l'obiettivo della CGIL: come è stato possibile che non sia stato fermato? Oggi sappiamo, per esempio, che la procura aveva chiesto ad agosto di arrestarlo per le continue violazioni degli obblighi imposti dalla sorveglianza. Abbiamo saputo anche che, però, il giudice aveva detto no. Ecco perché Castellino stava in quella piazza. Ma perché dopo averlo sentito dire «assediamo la CGIL» non è stato arrestato? E perché la sede della CGIL, obiettivo sensibile, non era ben presidiata dalle Forze dell'ordine per respingere l'assalto? Lei ha parlato, se non ricordo male, di 20 uomini davanti alla sede della CGIL e ce n'erano 1.500 tumultuosi, così li ha definiti nella sua informativa. Certamente, in quel contesto l'arresto in piazza dell'esponente di Forza Nuova avrebbe potuto provocare una reazione violenta; in quelle circostanze vale la regola della riduzione del danno, è vero, ma non possiamo non ribadire qui che l'assalto alla CGIL è stato un attacco alla nostra democrazia e alla nostra Costituzione, che è antifascista. La *leader* di Fratelli d'Italia ha sostenuto che ci sia una regia dello Stato che ci farebbe tornare agli anni bui, alla strategia della tensione, che Forza Nuova sia stata lasciata di proposito a briglia sciolta: è un goffo tentativo di depistaggio, un far caciara, come dicono a Roma. Noi, invece, stiamo sulla questione; noi esprimiamo solidarietà alle Forze di polizia. Riprendo un articolo di Paolo Berizzi, il giornalista di «la Repubblica» sotto scorta minacciato dai neofascisti: era il 10 ottobre di un anno fa - scrive Berizzi - quando i capi di Forza Nuova, insieme a no vax e no mask, diedero vita a un esecutivo che nei loro piani avrebbe dovuto sostituire il Governo Conte. Un'iniziativa che, riletta adesso, dopo la violenta azione eversiva del 9 ottobre, con l'attacco ai palazzi delle istituzioni e l'intenzione dei manifestanti no *green pass* di occupare Palazzo Chigi e Parlamento - come poi hanno fatto nella sede del primo sindacato italiano - suona quasi profetica, e comunque piuttosto inquietante. Per questo, ministra Lamorgese, le rinnovo la nostra solidarietà, chiedendole nello stesso tempo un cambio di passo. Bisogna garantire la libertà di manifestazione, ma non può esserci legittimità per i violenti e i fascisti di questo millennio. C'è un prima 9 ottobre e ci deve essere un dopo 9 ottobre: sottovalutare quei movimenti rappresenterebbe una tragica replica di momenti già vissuti e le nostre istituzioni non possono, non devono commettere simili errori di cui si porterebbero tutte le responsabilità. Viva la CGIL, viva il sindacato, viva l'Italia antifascista!

Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signora ministra Lamorgese, noi non le chiederemo le dimissioni, ma questo non ci esime dall'esprimere perplessità sulla gestione dell'ordine pubblico durante la fase finale

che hanno soffiato sul fuoco al punto da rendere protagoniste, loro malgrado, anche le Forze dell'ordine nella competizione elettorale. A quelle donne e a quegli uomini con la divisa va la nostra solidarietà; senza se e senza ma, noi siamo al vostro fianco, da Trieste, passando per Milano, sino alla sede della CGIL di Roma. Siamo al fianco di chi garantisce libertà e diritti di tutti, ma questo deve avvenire nell'alveo delle regole democratiche. Signora Ministra, mi permetta di dirle che, dinanzi a tanta solidarietà, auspico che alle parole seguano i fatti. Si dia luogo finalmente alla chiusura del contratto nazionale e si adeguino i mezzi in dotazione alle Forze dell'ordine. In sintesi, si diano le garanzie funzionali: oggi un carabiniere che va a processo non ha alcuna tutela legale e questo è sperequativo rispetto a ciò che accade ad altri servitori dello Stato. Nel merito della gestione, signora Ministra, ci sono state troppe falle precedenti alla manifestazione di Roma e troppe durante il suo svolgimento. C'erano solo sette agenti a difesa della sede della CGIL, nonostante gli annunci minacciosi di personaggi troppo noti da essere sottovalutati e persino liberi di circolare. Quelle immagini dei nostri poliziotti malmenati è una ferita che lede la dignità della nostra democrazia. *(Applausi)*. Si è trattato di un'aggressione non solo di neofascisti, ma anche di piccole frange che hanno abbandonato consapevolmente la protesta democratica per dare luogo ad atti criminali. La saggezza e il sangue freddo delle nostre Forze dell'ordine dinanzi a questa deriva di violenza hanno evitato che ci scappasse il morto. La politica non deve versare benzina sul fuoco, perché il rischio di un punto di non ritorno è dietro l'angolo. Attenzione, però, signora Ministra, a non catalogare con definizioni semplicistiche gli oltre tre milioni di lavoratori nostri concittadini che non si sono vaccinati, solo perché magari non credono nell'obbligatorietà del *green pass*. Le maglie larghe tra l'obbligo del *green pass* e la facoltà di vaccinarsi alimentano la narrazione di un Governo che agisce in modo pilatesco, ossia non si assume la responsabilità di rendere obbligatorio il vaccino. Lo voglio dire con chiarezza: noi rigettiamo queste tesi. Grazie ai vaccini e grazie al *green pass* l'Italia torna libera e torna a vivere, ma nove milioni di nostri concittadini non vaccinati chiedono a tutta la politica un *surplus* di analisi che non può essere archiviato con epiteti o con la messa al bando degli stessi protagonisti. In termini di legalità, mi permetta un'ultima considerazione non polemica, La manifestazione indetta dalla CGIL a San Giovanni nel sabato precedente le elezioni, quindi nel giorno del silenzio elettorale, crea un precedente, una deroga che neanche durante il periodo del terrorismo è stata posta in essere. Abbiamo aderito allo spirito della piazza contro ogni forma di violenza, ma perché non condannare anche gli atti violenti provenienti dall'estrema sinistra? Perché non condannare in quella piazza gli atti vandalici subiti dal comitato Michetti con la stella delle Brigate Rosse? Neanche una parola di condanna è arrivata da quella piazza. Troppo facilmente, nel nostro Paese, quando non si comprende, non si condivide o semplicemente non si apprezza, si ricorre a definizioni semplicistiche. Non esistono soluzioni o definizioni facili, sarebbe un solo *slogan* e noi non parleremo mai per *slogan*. Mi permetta di ricordare un giornalista (in tanti non hanno mai parlato per *slogan*, ma sono stati vittime dell'onta, quando hanno detto la verità): ricordo Giampaolo Pansa, che ha scritto il libro «Il sangue dei vinti»;

perché il rischio è che si vada fuori controllo e si generi un clima che riporta indietro le lancette del tempo, a cui noi non ci rassegneremo mai.

in Italia spesso la criminalità organizzata va cercata nelle prefetture. Oibò, da Ministro dell'interno, io avrei chiesto immediatamente o i nomi o le dimissioni. Sono passati dieci giorni.

e lascia che qualcuno che ricopre un incarico così importante affermi pubblicamente che nelle prefetture si annidano mafiosi e camorristi? Non è normale. Non è colpa dei fascisti: in questo non c'entrano Forza Nuova e i fascisti. È una questione che il Ministro dell'interno, che si occupa di pubblica sicurezza, e il Presidente della Commissione antimafia, che ricopre un ruolo importante, dovrebbero chiarire a codesto Senato, perché da cittadino italiano, se nella mia prefettura di riferimento (quella di Milano) si annidano dei mafiosi, vorrei saperlo: quindi uno dei due

se sui banchi del Governo ci fosse stato il ministro Salvini: il ministro Salvini ha permesso che dei fascisti, che non potevano essere in piazza, annunciassero l'assedio alla CGIL e poi ha ordinato ai poliziotti di non intervenire, permettendo dopo un'ora e mezza l'assedio alla CGIL. Amici del

se qualcuno ai massimi livelli fa bene il suo lavoro, onore al merito. Appositamente non parlo degli sbarchi, dei rimpatri, delle *baby gang*: ne stanno succedendo di tutti i colori. Parlo di quello che è accaduto settimana scorsa, che ci ha fatto fare una figura meschina a livello mondiale. Signor Ministro, si prenda le sue responsabilità. Se non ha capito che cosa stava succedendo, è grave. Se l'ha capito e l'ha permesso, è ancora più grave. È molto semplice. Se il Sottosegretario con la delega ai Servizi non è in grado di stabilire se in una piazza arrivano 1.000 o 15.000 persone, è un problema.

su cui rispondere e non possono essere le 10, 20 o 30 pagine scritte con amore da solerti funzionari pubblici - le scrivevano a far passare in secondo piano quella che è stata una *débâcle*: 41 poliziotti feriti non sta né in cielo, né in terra. Signor Ministro, chieda aiuto a quest'Assemblea, a qualcuno che le può dare una mano; non viva con insofferenza la presenza del Parlamento. Non si isoli nei suoi uffici, perché purtroppo ci sono questori e prefetti che si sentono soli; ci sono dirigenti delle questure che si sentono soli; ci sono poliziotti che, se non sono tutelati dal massimo vertice della pubblica sicurezza, fanno il loro lavoro con uno spirito diverso. Se ci sono poliziotti isolati,

Sì, è una vergogna, è vero, perché abbiamo parlato per dieci giorni dell'emergenza fascista, mentre l'emergenza di questo Paese è il lavoro, lavoro e ancora lavoro. Se non riuscite a isolare venti imbecilli, che tutti conoscono per nome e cognome, vuol dire che non sapete fare il vostro mestiere. Non sono sbarcati da Marte; uno di loro ha il braccialetto elettronico e il Daspo per non andare a vedere la Roma, tuttavia arringava 10.000 persone in Piazza del Popolo. Se uno vuole andare allo stadio senza il *green pass*, lo portate fuori per le orecchie e tuttavia permettete che questi delinquenti mettano a ferro e fuoco una città. C'è qualcosa che non funziona, ma non abbiamo sentito una sola parola di autocritica su questo. *(Applausi)*. Speriamo che non succeda più. Quando arriveranno Biden e gli altri *leader* del mondo, spero che non ci siano quest'approssimazione, questa sciatteria e quest'inadeguatezza, perché non ce le possiamo permettere. La gente si aspetta certezza in questo momento. Certo, chi fa il suo lavoro può sbagliare, per carità di Dio; però a me piacciono quelli che si prendono le responsabilità

ci vado orgoglioso di quello che ho fatto da Ministro dell'interno, perché ho scelto di non voltarmi dall'altra parte. Dopo il Covid, penso che questo ruolo sia ancora più delicato, quindi, signor Ministro, le do un consiglio: faccia sentire la sua vicinanza a chi lavora non sotto di lei, ma di fianco a lei. Mai dire: chiedete al prefetto, chiedete al questore, chiedete al funzionario, chiedete al responsabile dell'ordine pubblico di quella piazza. Ma vi pare normale che ci sia stata una manifestazione di parte e di partito il sabato prima del voto a Roma e che ci siano stati lacrimogeni e idranti lunedì con le urne aperte a Trieste? *(Applausi).* Neanche in Cile e in Venezuela,

di ascoltare; però, a parti invertite, avreste chiesto l'invio dei caschi blu dell'ONU. Non so se vi rendete conto dell'ipocrisia che alberga a sinistra, della profonda ipocrisia che alberga a casa vostra. *(Applausi).* Abbiate almeno Buon lavoro, signor Ministro, se comincerà a fare il Ministro, perché per il momento non ce ne siamo ancora accorti.

ringrazio la signora Ministra per il suo necessario intervento. Onorevoli colleghi, le immagini dell'assalto alla sede nazionale della CGIL e degli scontri con le Forze dell'ordine avvenuti a Trieste, a Milano centro di Roma non possono lasciare nessuno di noi indifferente. Il diritto di manifestare le proprie idee non può mai degenerare in atti di aggressione, intimidazione e violenza. I valori dell'antifascismo e della resistenza e il ripudio dell'ideologia autoritaria rappresentano il fondamento della nostra Costituzione, nata da un accordo trasversale tra forze politiche diverse, basata su principi espressi sia nella XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, che vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista, sia nella relativa disposizione di attuazione prevista dalla cosiddetta legge Scelba, che ha recepito in pieno questa norma. Detto precetto costituzionale, fissando un'impossibilità giuridica assoluta e incondizionata, impedisce che un movimento formatosi e operante in violazione di tale divieto possa in qualsiasi forma partecipare alla vita politica e condizionarne le libere e democratiche dinamiche. Gli avvenimenti di sabato 9 ottobre, culminati con l'efferato attacco rivolto alla più antica organizzazione sindacale italiana, la CGIL, rappresentano un autentico attentato alla democrazia del nostro Paese, rammentando che i sindacati sono espressione di libertà e tutela della dignità del lavoratore. Quanto accaduto deve imporre a noi tutti una profonda riflessione: risulta necessario e non più rinviabile un forte e decisivo intervento nel fronteggiare un fenomeno sempre più pericoloso e troppo a lungo sottovalutato, ridotto a banale folklore. Occorre programmare in maniera precisa e puntuale le misure di sicurezza da adottare, al fine di prevenire questi drammatici eventi, coinvolgendo tutte le Forze dell'ordine, in modo da evitare che sia messa in pericolo l'incolumità pubblica, ma soprattutto quella dei singoli poliziotti, presenti per motivi di lavoro, e degli stessi manifestanti pacifici, anche con l'ausilio di strumenti tecnologici innovativi. Un ringraziamento va alle Forze dell'ordine, che spesso si trovano a dover fronteggiare situazioni critiche con scarsità di mezzi, al personale sanitario, eroe di questa pandemia. Occorre usare senza rinvii la legislazione esistente, per sciogliere finalmente le formazioni che si ispirano alla cultura e alla storia fascista e nazista; occorre dare impulso alla conoscenza del fascismo, delle sue origini e della tragedia che ha rappresentato insieme al nazismo, dando rinnovato vigore alle radici e allo spirito della nostra Costituzione, Costituzione, divulgando tali principi in tutte le sedi e in tutte le istituzioni, iniziando dalle scuole. Occorre con determinazione avere il coraggio di denunciare questa cultura basata sull'odio, sulla discriminazione, sull'intolleranza e sul razzismo, che soffia sul disagio sociale e lo strumentalizza. *(Applausi)*. Occorre tessere nuovamente i fili di una regolare partecipazione democratica, per operare un'organica ricostruzione del Paese, basata sui valori costituzionali, per i quali i nostri Padri costituenti hanno combattuto, per un'idea di *res publica* elevata, scevri da qualsiasi tornaconto elettorale, ricostruendo un'efficace rete di diritti e tutele universali, ridando dignità al lavoro umiliato, frammentato e diviso. Nessuna libertà di pensiero dev'essere adottata a giustificazione di quanto avvenuto. Per questo, signora Ministra, invito lei e tutte le forze politiche presenti in quest'Aula a perseguire quanto disposto dal dettato costituzionale, adottando tutti i provvedimenti necessari per assicurare livelli maggiori di sicurezza, implementando le Forze dell'ordine esistenti sul territorio

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 28 ottobre. L'ordine del giorno della seduta di domani, alle ore 9, prevede le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre 2021. A partire dalle ore 14,30, saranno discusse mozioni su iniziative volte a dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e mozioni su iniziative volte a contrastare ogni forma di violenza e di totalitarismo. La discussione delle mozioni potrà proseguire, ove necessario, nella seduta di giovedì 21 ottobre. Martedì 26 ottobre, a partire dalle ore 16,30, avrà luogo la discussione del decreto-legge sugli incendi boschivi. La seduta non prevede orario di chiusura. Il calendario della prossima settimana prevede inoltre i seguenti argomenti: il seguito della discussione del disegno di legge sul contrasto della discriminazione e violenza per sesso, genere e disabilità, approvato dalla Camera dei deputati; la legge europea 2019-2020, già approvata dalla Camera dei deputati, e connesse relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea; il disegno di legge, collegato alla manovra di bilancio, già approvato dalla Camera dei deputati, sui titoli universitari abilitanti; la prima deliberazione del Senato sul disegno di legge costituzionale di modifica all'articolo 119 della Costituzione per il riconoscimento dello svantaggio derivante dall'insularità.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

la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esso correlati, in data 24 marzo 2021, ha approvato all'unanimità la relazione sull'inquinamento derivante dall'utilizzo dei gessi rossi prodotti a Scarlino, Comune di Grosseto, in Toscana, quella Toscana dove da anni i presidenti regionali, coloro che dovrebbero tutelare il bene comune, sono politici del La relazione dovrebbe essere dibattuta in quest'Aula. In sette mesi, però, un argomento così delicato ed evidentemente di appartenenza politica non ha trovato spazio. In quel luogo e in quella Regione ci sono vergognosi guadagni sulle spalle della gente. Dalla relazione emerge infatti un risparmio illecito di ben 237 milioni a fronte di uno sfrontato e accertato inquinamento delle falde acquifere. Perché allora rimandare un argomento così importante, studiato, valutato e condannato da una Commissione il cui ruolo è così svalutato e soprattutto subordinato ai poteri forti di una parte politica? Si parla in continuazione di *green* e poi sull'inquinamento delle falde acquifere si china il capo davanti al dio denaro; troppa ipocrisia e furbizia politica. Mi chiedo a questo punto utile il ruolo della Commissione e segnalo comunque la necessità che arrivi in Aula la discussione sui gessi rossi, soprattutto ora che le elezioni sono concluse. Chiudo leggendo le conclusioni oggettive e coraggiose della Commissione: non pare che questo sia l'atteggiamento corretto da tenere da parte dello Stato e delle Istituzioni pubbliche che dovrebbero tutelare l'ambiente. Più correttamente, la soluzione che si sarebbe dovuta adottare era quella di vietare l'uso dei gessi per il ripristino delle ex cave cave esaurite. Vado oltre, perché la relazione conclude con una frase che schiaffeggia la politica: «Trovato l'inquinamento, la legge lo mantiene». Rinnovo la necessità di portare in Aula questo argomento, che evidentemente interessa il PD.

per ricordare, prima di tutto a me stesso, la figura di una persona che ieri ci ha lasciato, un sardo che nella sua estrema umiltà ha dato lustro alla Sardegna, guadagnandosi l'appellativo di eroe, che però ha sempre rifiutato. Parlo di Angelo Licheri, l'uomo che, mettendo a repentaglio la propria vita in maniera del tutto gratuita e generosa, aveva tentato di salvare Alfredino Rampi in quelle terribili giornate che a noi tutti sono note e serbiamo nel nostro ricordo. Angelo Licheri era una persona molto umile, provata nel fisico, senza una gamba a causa del diabete, semicieco e con gravi problemi all'udito. In tutto questo, comunque, continuava a mantenere vivo il ricordo di quella notte e ad avere il coraggio del rifiuto, pur vivendo nell'estrema indigenza: gli avevano gli avevano offerto 27 medaglie d'oro, ma consapevole - diceva lui - di aver fallito in quell'impresa assolutamente difficile, ha sempre rifiutato. Ho inteso parlare perché qualche mese fa, assieme al presidente Faraone, abbiamo presentato una mozione per fare in modo che quest'uomo potesse almeno avere la dignità di una vita serena e di un fine vita sereno, perché gli era stato rifiutato qualsiasi tipo di aiuto e viveva davvero nell'indigenza, ospite di una casa di riposo. Purtroppo quella mozione non è mai stata portata all'esame dell'Assemblea e non è mai stata discussa. Quest'uomo diceva di essere ricordato soltanto nei giorni dell'anniversario della vicenda di Vermicino e lamentava di non aver mai gli auguri, neanche a Natale né a Pasqua; in questo senso, a me rimane il rimorso di non essere riuscito a portare a termine quell'operazione e credo che su questo dovremmo riflettere, perché abbiamo davvero tante figure come Angelo Licheri, che però forse non valorizziamo, non ricordiamo e non aiutiamo abbastanza. Salutiamo quindi anche da quest'Aula, con la solennità che quest'Assemblea merita, la figura di un eroe che ha davvero messo a repentaglio la sua vita in maniera gratuita, semplicemente nel tentativo di salvarne un'altra.

onorevoli colleghi, il mio intervento vuole porre l'attenzione su una realtà estremamente positiva, che rappresenta un successo per i nostri scienziati e le professionalità presenti nel nostro Paese, in particolare, in questo caso specifico, nella mia Regione, la Campania. Vi sono figure di alto profilo nel panorama scientifico e nella ricerca mondiale che confermano ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, le enormi potenzialità e le grandi competenze della nostra ricerca e dei nostri ricercatori.

In particolare, in questo caso, dieci bambini hanno ritrovato la vista grazie a una terapia genica, eseguita per la prima volta in Italia nell'azienda ospedaliera dell'Università degli I piccoli erano ipovedenti a causa di una rara forma di distrofia retinica ereditaria legata a mutazioni genetiche. Il risultato ottenuto è il frutto del lavoro certosino e approfondito condotto dalla clinica oculistica universitaria in collaborazione con Telethon e il Children's Hospital di Philadelphia. I bambini non erano campani e provenivano da diverse Regioni italiane. Vorrei fare una considerazione importante: Napoli diventa punto di riferimento nazionale per il trattamento di malattie rare della retina. Non più quindi solo viaggi della speranza e di emigrazione sanitaria verso le Regioni centro-settentrionali, più organizzate e strutturate dal punto di vista sanitario, capaci di rispondere in maniera più appropriata e veloce alla domanda di salute di cittadini del Sud, le cui Regioni pagano anni di malasanità, carenze strutturali e organizzative e di piante organiche inadeguate. I dieci pazienti trattati oggi possono scrivere, leggere e muoversi in autonomia; la via del trattamento precoce in una patologia degenerativa come questa è fondamentale. Il successo, frutto di anni di lavoro e di ricerca, permette di offrire una speranza reale di vita migliore ai piccoli pazienti. Occorre essere orgogliosi del *team* di ricerca che ha ottenuto questo grande risultato, che pone il nostro Paese all'avanguardia in Europa.